interrogato su questa vicenda che riguarda il territorio del quale entrambi siamo stati espressioni come collegio elettorale e al quale ci sentiamo profondamente legati, ha lodevolmente e naturalmente fatto affidamento sull'imparzialità e sul lavoro senz'altro encomiabile della magistratura, al quale naturalmente mi sono associato e continuo ad associarmi anch'io da garantista non dell'ultima ora, ma, venendo evidentemente frainteso dalla stampa, anche sottolineato che in quel Comune si è lavorato comunque bene. Credo che tale espressione sia stata letta dai *mass media* in maniera errata e strumentale; senz'altro essa non voleva, in alcun modo, suonare come un'attenuante o una scusante di atteggiamenti poco commendevoli, ma, purtroppo, la stampa ha riportato la notizia che generano questo dato e vi è stata anche una polemica tra le forze politiche. Siccome sono convintissimo e lei sarà convinto quanto me

Ci prepariamo a discutere un atto importante, cioè il decreto collegato alla manovra finanziaria.

L'attuale maggioranza è capace di andare avanti - e non voglio aprire una polemica - anche senza il contributo dei senatori a vita, perché spesso si può votare con meno parlamentari; c'è una battaglia politica, però, santo cielo, lei, in una delle ultime sedute, quando tale questione fu sollevata, ebbe il garbo di dire che avrebbe fatto di tutto, senza interferire nell'attività dell'Esecutivo, per far capire al Governo che il Parlamento è sovrano e deve poter discutere.

si è deciso, rispetto alla pregiudiziale, di ignorare gli elementi di evidente incostituzionalità riconosciuti anche dalla 1a Commissione. Signor Presidente, la prego di fare ogni sforzo possibile per convincere il Governo che siamo ancora in una democrazia in cui il Parlamento ha il diritto di essere rispettato. Signor Presidente, ho chiesto di poter intervenire sull'ordine dei lavori per sottolineare una vicenda incresciosa che è si è verificata qualche giorno fa,

Ministro ha affermato, in un modo a dir poco vergognoso, che la storia della Democrazia Cristiana è stata segnata, in un particolare momento

e che tutto il resto della storia della Democrazia Cristiana è stata storia di delinquenti e di persone da mettere in galera. Signor Presidente, le rivolgo una protesta formale perché la storia della Democrazia Cristiana non la può intestare sicuramente un ex magistrato, ora ministro della Repubblica, come l'onorevole Di Pietro.

noto negli ambienti di piazza del Gesù, almeno in quel periodo, sia stato anche lui complice e abbia comunque messo il cappello su dichiarazioni irresponsabili del ministro Di Pietro.

che le agenzie di stampa stanno battendo questa mattina relativamente ad un episodio apparentemente minore ma, a mio giudizio, comunque preoccupante che si sta verificando nel nostro Paese.

al sequestro di bussole radioattive contenenti radio 226. Si tratta di una sostanza fortemente radiotossica che nel secolo scorso (nel 1900) veniva usata, come precisano peraltro le agenzie, nell'attività dei poli oncologici per la cura dei tumori in brachiterapia ed anche in alcune lavorazioni di vernici poi abbandonate. Si deve pertanto ritenere che i prodotti che vengono sequestrati e che sembra siano commercializzati in negozi di articoli militari come se niente fosse debbano provenire dal residuo di sostanze lavorate negli ospedali o altrove in anni passati. Signor Presidente, la Commissione bicamerale d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti, della quale ho avuto da lei l'onore di essere chiamato a far parte, sicuramente affronterà, una volta insediata, questo problema, che però, mi pare di capire, può suscitare qualche allarme nell'opinione pubblica. Teniamo conto che secondo le notizie questi sequestri sono già avvenuti a Torino, Bologna, Udine, Firenze, Ancona e in altre località del nostro Paese. Mi sembra opportuno sottolineare che, fermo restando che non bisogna dare più allarme di quello che c'è, si tratta di notizie preoccupanti che richiedono attenzione ed è bene che anche il Parlamento nelle forme dovute - mi riservo di presentare atti ispettivi al riguardo - se ne faccia carico.

un giudizio politico altrettanto laconico: mi pare però che, al di là dei fatti citati, le amministrazioni che si sono succedute hanno anche cambiato positivamente il volto della città. Queste sono le due affermazioni, non

la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ha approvato all'unanimità il calendario dei lavori dell'Assemblea fino al 21 dicembre. In mattinata è confermato il prosieguo della discussione generale sul decreto-legge collegato in materia fiscale. Oggi pomeriggio, dalle ore 16,30 alle ore 17,30, quindi per un'ora, riprenderanno le votazioni sui restanti articoli ed emendamenti al disegno di legge comunitaria, nell'auspicio di concluderne la trattazione in tale lasso di tempo. Proseguirà quindi la discussione generale del decreto-legge collegato fino alle ore 21. Le repliche dei relatori e del Governo avranno luogo nella seduta antimeridiana di domani. A conclusione di tale seduta, sarà data lettura della comunicazione del Presidente ai sensi dell'articolo 126, comma 4, del Regolamento, sul contenuto del disegno di legge finanziaria. Da quel momento avrà formale inizio la sessione di bilancio. Le Commissioni permanenti comunicheranno entro le ore 13 di mercoledì 29 novembre i propri rapporti sui documenti di bilancio alla 5a Commissione permanente, che concluderà l'esame di propria competenza entro sabato 9 dicembre. Gli emendamenti per l'Assemblea dovranno essere presentati entro le ore 12 di domenica 10 dicembre. Nel periodo dal 27 novembre al 9 dicembre l'Assemblea non terrà seduta per consentire alla 5a Commissione permanente un esame approfondito dei documenti di bilancio.

Ricordo infine che il calendario della settimana corrente prevede i documenti definiti dalla Giunta competente in materia di insindacabilità e l'esame della riforma dell'articolo 5 del Regolamento del Senato,

Presidente, intervengo per porle una questione che credo riguardi la sovranità dell'Assemblea e il ruolo che lei stesso è chiamato a svolgere come oggi un quotidiano nazionale sottolineava rispetto al tema della fiducia, è una sorta di ruolo pedagogico. Un tentativo di fare pedagogia istituzionale che tuttavia rischia di non concretizzarsi con la possibilità per il Parlamento, in questo caso il Senato, di svolgere la sua funzione.

Il Ministro, ad un certo punto della sua riflessione, dice chiaramente che sarà inevitabile

della fiducia annunciata a mezzo stampa e, addirittura, in via preventiva rispetto all'avvio della sessione di bilancio di cui lei ha parlato poco fa.

con il meccanismo del maxiemendamento si instaura una prassi in base alla quale la compensazione, la contrattazione e il punto di equilibrio

la sintesi e determina le condizioni per prospettare al Parlamento la blindatura del pacchetto chiuso del maxiemendamento. Lo stesso Presidente della Commissione bilancio - che non vedo in Aula

alla fine del dibattito in Commissione, che è un tentativo comprensibile di coniugare le esigenze di velocizzazione dei tempi di approvazione con il rispetto della dialettica e del dibattito parlamentare. Presidente, è grave che un Ministro - soprattutto il Ministro per l'attuazione del programma - prima ancora che inizi la discussione della sessione di bilancio

Parlamento, e di perpetuarne l'immagine come un pedagogo delle istituzioni, che, tuttavia, nella prassi e nella pratica, non riesce - come pure sicuramente vorrebbe - a tutelare la sovranità e la dialettica parlamentare come elementi fecondi di discussione, di dibattito, di qualità della politica e di capacità di esprimere l'alternatività rispetto allo strumento fondamentale della legge finanziaria dello Stato.

è molto importante, perché - com'è già stato ricordato - assicura una quota significativa delle risorse per la copertura della manovra di bilancio e costituisce, quindi, l'avvio, sia pure non formale, della nostra sessione di bilancio. Lei ha testé annunciato, signor Presidente, il calendario di tale sessione,

Vorrei rivendicare preliminarmente - farò brevi considerazioni a nome del Gruppo dell'Ulivo - il metodo che abbiamo seguito nella discussione del provvedimento. di una rivendicazione che ha a che fare con la questione posta poco fa e su cui lei, signor Presidente, ha giustamente fatto un rinvio al dibattito e al modo in cui si organizzano i lavori in vista della legge finanziaria in Commissione bilancio. bilancio. Voglio rivendicare la trasparenza dei comportamenti della maggioranza in Commissione e l'approfondito dibattito che si è svolto in quella sede su questo provvedimento. la trasparenza, abbiamo annunciato, fin dall'inizio della discussione sul decreto-legge, che non avevamo intenzione di apportare modifiche allo stesso e che, in parte per evitare ingorghi parlamentari e sovrapposizione di questa discussione con il dibattito sulla legge finanziaria e, in parte per dare un segnale preciso

detto e - mi pare - mantenuto che non per questo intendevamo fare una discussione meno seria. In effetti, discussione seria c'è stata: abbiamo approfondito i punti principali; come hanno ricordato i relatori, abbiamo individuato nel dibattito questioni che anche nella valutazione della maggioranza meritano un approfondimento e che siamo pronti a discutere e a modificare nella legge finanziaria.

il tema delle auto aziendali, il tema delle norme in materia di catasto, il tema delle concessioni autostradali, il tema delle norme in materia di enti di ricerca. Sono questi i titoli principali di un ragionamento che la maggioranza ha fatto in Commissione in ordine alla necessità di un approfondimento e questo ragionamento lo ha svolto non da sola, ma insieme con l'opposizione. Do atto volentieri all'opposizione di aver offerto un contributo significativo alla discussione in Commissione bilancio e di aver interloquito soprattutto su questi temi - ma anche su altri - positivamente. Credo che le decisioni che abbiamo preso e gli orientamenti che abbiamo espresso abbiano in qualche modo a che fare anche con la discussione che

Allora, come lei ricordava, signor Presidente, non è banale immaginare che la Commissione è un luogo importante del confronto parlamentare sulla manovra di bilancio.

che conduca a modificazioni, impegni, ragionamenti comuni, come abbiamo fatto sul decreto e come faremo sulla legge finanziaria. Quindi, ci sentiamo di dire che è pienamente assicurato, attraverso questo metodo, il dibattito e il confronto parlamentare sugli elementi principali della manovra di bilancio. signor Presidente, proprio da questo confronto emergono le differenze. Sono emerse differenze significative in ordine alla strategia, anche di politica economica. Ne ricordo soprattutto una. Ho dato una scorsa

che ci ha impegnati a lungo: la strategia che abbiamo collocato nel decreto, che per noi costituisce un elemento fondamentale per completare la strategia di lotta all'evasione fiscale, iniziata con il decreto di luglio per reperire risorse, ma anche per impostare una nuova cultura nel rapporto tra l'amministrazione fiscale e il contribuente che crei una situazione di normalità, che superi quel dato paradossale e - l'hanno ricordato i relatori molto bene e meglio di quanto posso fare io

Ebbene, su questo si sono manifestate le differenze perché l'opposizione ha proposto emendamenti soppressivi di tutte le norme relative alla lotta all'evasione fiscale, sostituendole con tagli orizzontali ai capitoli di bilancio.

Pertanto, non esiste un'ipotesi di reperimento di risorse basata semplicemente sulle operazioni inerenti al bilancio. Siamo convinti che una strategia seria di lotta all'evasione fiscale sia la premessa

Come hanno ricordato i relatori, all'articolo 1 della legge finanziaria introdurremo una norma che prevede di destinare a riduzione delle aliquote le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale.

sul tema della strategia di politica economica da mettere in campo, facendo riferimento alle tre critiche fondamentali che sono state rivolte alla manovra.

La strategia dello sviluppo è la strategia della nostra legge finanziaria ed oggi iniziamo un percorso che ci condurrà ad approvare provvedimenti importanti per la crescita ed il futuro del nostro Paese.

Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, dopo l'onesta difesa d'ufficio del collega Morgando (che rispetto per averlo conosciuto in tutta la sua correttezza in Commissione bilancio alla Camera, nella scorsa legislatura),

Comunista, che ha tracciato la linea, che diceva: «Anche i ricchi piangano». Ebbene, si è dato corso ad una manovra finanziaria, di cui questo decreto è parte importante, che obiettivamente non era necessaria. Una manovra da 34 miliardi di euro,

stati sufficienti. Rispetto a quanto sta avvenendo in Europa, dove si cerca di ridurre la pressione fiscale, tagliare e razionalizzare lo Stato sociale e l'intervento del pubblico nell'economia, nella nostra manovra finanziaria finanziaria sta avvenendo l'esatto contrario. Stiamo assistendo ad una manovra che porta la pressione fiscale ai livelli maggiori d'Europa (43 per cento); siamo in controtendenza su tutto, come sempre. La manovra era partita impostata su una linea che potremmo definire da novelli Robin Hood: «togliere ai ricchi per dare ai poveri».

fossero dei grandi capitalisti, non sapendo che invece, in Italia, la gran massa è su livelli piccoli e medi. Vengono rivalutate le rendite catastali, fondamentali per l'individuazione dell'ICI, del 40 vengono modificate, per citare altri attacchi a chi produce e a chi lavora, le quote di ammortamento deducibili per fabbricati e macchine strumentali dell'impresa, con oneri aggiuntivi del 30

della carta moneta. In questo modo si avrebbe sicuramente il controllo di ogni transazione finanziaria e non ci sarebbero più elusione ed evasione fiscale. Poi vi lamentate se già tutti stanno cercando di correre ai ripari e probabilmente nelle prossime dichiarazioni dei redditi o iniziative o iniziative fiscali che ci saranno nel nostro Paese ci sarà un aumento dell'evasione! Cosa volete che facciano un piccolo imprenditore o un lavoratore che ha delle integrazioni con altri redditi di fronte al fatto che che non date niente in contropartita a queste nuove imposizioni, anzi assumete ben 300.000 precari nella pubblica amministrazione senza introdurre criteri di efficienza e di produttività? per cui, come dicevo, siete passati da un provvedimento di natura classista a uno di natura interclassista, é che alla fine andrete a colpire profondamente soprattutto gli operai ed i pensionati, perché i trasferimenti a copertura dei minori trasferimenti alle Regioni e ai

per colpire i ricchi e farli piangere e alla fine fate piangere tutti, oppure siete dei dilettanti allo sbaraglio. Penso che questa finanziaria e questo provvedimento vedano l'intero Paese contro di voi: il 70 per cento del Paese è contro di voi, lo attestano le indagini demoscopiche e le manifestazioni di massa. Credo che il segnale che arriva dal Paese

dell'attuale coalizione, comincino i ragionamenti per il superamento dell'attuale Governo Prodi. È impossibile che questo nostro Paese vada avanti ancora in questa direzione: rischiamo di avere non un Paese impazzito, ma un Paese talmente sfiduciato da non avere alcun tipo di voglia di fare e profondamente demotivato.

State facendo dei capolavori formidabili. Mi auguro, e concludo, che questo provvedimento - che aveva l'obbiettivo di far piangere i ricchi e alla fine farà piangere anche i poveri - sia l'ultimo provvedimento dannoso del Governo Prodi e che dall'inizio del prossimo anno si aprano una nuova prospettiva e un nuovo scenario politico per questo nostro Paese. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento in discussione, collegato alla legge finanziaria, con la quale costituisce un *unicum,* contrariamente a quanto è stato detto dal Governo, non ha aiutato e non aiuterà la crescita del Paese. Da mesi non solo l'Italia produttiva, e cioè le imprese e le professioni, ma anche i più autorevoli economisti hanno lanciato l'allarme sul clima di sfiducia che proprio grazie a questi provvedimenti l'opinione pubblica ha verso il Governo e le istituzioni. Diceva qualche tempo fa l'opinionista Sergio Romano: «non credo vi sia stato un altro momento politico in cui i sentimenti di stima e fiducia della società per il vertice del Paese soprattutto politico ma anche economico abbiano toccato un punto così basso». La ragione di tutto ciò è il modo ideologico in cui è stata concepita la manovra economica e il suo strumento propedeutico in discussione questa mattina, cioè il cosiddetto decreto fiscale, dove le misure per lo sviluppo sono inesistenti o si sono confermate, come nel caso delle cosiddette liberalizzazioni, semplicemente dei palliativi. Infatti, il Governo ha in testa un'unica cosa: tenere buona l'ala massimalista della sua compagine e quindi - come ha fatto - aumentare la pressione fiscale ed, anziché contenere la spesa pubblica, aprire i cordoni della borsa per accontentare coloro che rivendicano diritti credendo, in questo modo, di centrare l'obiettivo della redistribuzione del reddito. Con questo atteggiamento, Prodi alimenta peraltro uno dei sentimenti più perversi della nostra società e cioè la rivendicazione dei diritti anziché la cultura dei doveri. Se l'equità sociale è un obiettivo, infatti, l'egualitarismo è il contrario dello sviluppo e della crescita perché è soltanto l'appiattimento verso il basso di qualsiasi azione economica e sociale. D'altra parte, il Governo Prodi, fin dall'inizio, ha rinunciato alle riforme e scatenato la divisione sociale con una campagna di odio plasticamente raffigurata dallo slogan: «Anche i ricchi piangano», e si è poi impiccato al patto stupido europeo, così come era stato definito dallo stesso Prodi. in tutto il mondo, dall'America di Bush, che riduce le tasse ed è riuscita a generare in questo modo una robusta crescita (per cui dopo qualche anno di deficit al 4 per cento ora il *deficit* federale si avvia al 2 per alla Francia di Sarkozy, che ha già annunciato nel suo programma elettorale per le presidenziali del 2007 che privilegerà lo sviluppo piuttosto che il rispetto aritmetico dei parametri di Mastricht. L'errore di questo Governo è di non capire che il vero problema dell'Italia è innanzitutto la crescita e che essa può essere raggiunta solo creando fiducia nei cittadini e soprattutto fornendo loro maggiori risorse attraverso la leva fiscale, ovvero riducendo e non aumentando le tasse. Queste sono le condizioni generali, ma certamente non può essere trascurato il fatto che all'interno di esse diventano, ai fini dello sviluppo, determinanti le scelte sbagliate che il Governo ha fatto nei confronti delle attività produttive. infatti, non sono solo le tasse o i contributi previdenziali in senso astratto, come è evidente, ma è capire come esse incideranno sulla quotidianità. Ad esempio, ridurre il cuneo fiscale e bloccare le opere pubbliche è un errore. Il costo del lavoro, infatti, pur essendo in Italia fra i più elevati di Europa, non è la vera ragione della perdita di concorrenza delle imprese sui mercati internazionali; molto più incisiva sulla perdita di competitività delle aziende è la mancanza di infrastrutture dell'Italia. Un sano realismo avrebbe dovuto indurre il Presidente del Consiglio ad ascoltare anche le voci a lui più vicine e ricordarsi che prima di tutto, per rilanciare lo sviluppo, è necessario, come ha ricordato Bazzoli, presidente di Intesa-San Paolo, amico di Prodi, rilanciare le infrastrutture, fare un grande progetto. precedente Governo aveva tentato, fra le tante difficoltà, di fare del progetto di infrastrutturazione dell'Italia il perno e l'obiettivo della manovra economica e di sviluppo del Paese. Sono contento che gli amministratori della sinistra del Nord la pensino come me. Mi fa piacere leggere che il presidente Illy sostiene che i Presidenti delle Regioni settentrionali impiegherebbero un attimo a scrivere un documento comune contro il trasferimento forzoso del TFR allo Stato o contro l'aumento delle imposte, a prescindere dalle appartenenze politiche, e che il centro-sinistra si è giocato metà della sua credibilità omettendo nel programma la realizzazione della linea ad alta capacità e alta velocità che va da Lione a Trieste e arriva fino al confine ucraino: una linea che taglia tutto il Nord. Ora, il ministro delle infrastrutture Antonio di Pietro ha detto che la vuole realizzare - ha stabilito anche il termine - ma basta il voto contrario di un senatore di Rifondazione Comunista per far saltare tutto. A sinistra c'è chi sostiene che la TAV non serve e che basterebbe migliorare le vecchie linee. Non scherziamo! Illy dice che avrebbe messo nel programma anche la realizzazione del Ponte sullo Stretto. Ho riportato quasi per intero questa testimonianza perché è emblematica; in essa è scritto ciò che il Governo Berlusconi stava facendo ed è stato fermato. Aver bloccato questa azione significa aver impedito lo sviluppo dell'Italia ed aver abbassato la qualità di vita degli italiani. Termino con due esempi. Il vantaggio per le imprese di abbassare il cuneo fiscale costa allo Stato quest'anno - è scritto così in finanziaria - circa 2,5 miliardi di euro.

la mancanza di infrastrutture per le imprese italiane è valutata fra l'1,5 e il 2 per cento del PIL, cioè oltre 20 miliardi di euro. Questi aridi numeri servono a spiegare come ogni anno gravino sulle famiglie italiane e sulle imprese oltre 33 miliardi di euro di costi per mancanza di infrastrutture, cioè l'ammontare dell'intera finanziaria.... E' per questo che, a fronte di una modesta quanto relativa azione in favore delle imprese, il Governo non risponde al problema più vero dei cittadini e delle aziende, che è la modernizzazione del Paese. Da qui bisognava ripartire per dare un futuro al Paese. Questa del decreto fiscale e della finanziaria è un'occasione perduta. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento collegato alla manovra finanziaria non dovrebbe turbare né il popolo italiano, né il sistema produttivo, né il Parlamento, né le associazioni di categoria, per quanto esso abbia carattere di ripetitività ed abbia frequenza e cadenza annuali. Essersi verificato ciò che è accaduto, e cioè che tutto il mondo si sia lamentato di questo provvedimento legislativo, è la prova provata che evidentemente esso è dannoso, direi scellerato. Le motivazioni sono le seguenti. Si dice che la manovra fiscale e quella creditizia fossero strumenti nelle mani dei governanti per poter stimolare il sistema produttivo.

leva significa alleggerire, rendere meno pesante, consentire insomma al sistema produttivo di navigare in modo più accelerato e più efficace. Questo provvedimento collegato alla finanziaria

che, essendo così numerose, non possono non rivelarsi una vera e propria indebita agopuntura sul sistema produttivo italiano. Sono 67: è evidente che avrebbero generato una situazione di disagio globale. Cosa si sarebbe potuto fare per evitarlo? È presto detto. Noi con i nostri emendamenti riproposti anche suggeriamo un recupero di risorse riducendo la spesa corrente. Non inventiamo nulla, diciamo soltanto quello che la Banca d'Italia, inascoltata dal 1990 fino all'avvento del Governo Berlusconi, ha ripetuto:

Un Governo di sinistra-centro (dico volutamente di sinistra-centro perché dire di centro-sinistra sarebbe improprio), un Governo nel quale la sinistra è determinante, per quanto lo è con questo Governo, non può non pretendere di praticare politiche di sinistra sinistra esageratamente mirate. Ma noi sappiamo che nel tempo quelle politiche hanno portato all'impoverimento, all'attuazione della lotta di classe, hanno portato risultati non certamente utili né per l'umanità in generale, né per i Paesi laddove i Governi le hanno praticate. Avremmo voluto contenere, così come stavamo facendo, dando peraltro con una norma oltremodo virtuosa che avevamo preso a prestito da altro Paese europeo d'avanguardia, una elasticità nella spesa pari al 2 che aveva una funzione molto virtuosa, quella di cominciare ad abituare l'amministratore ad essere tale e non essere o considerarsi esclusivamente erogatore di spesa, perché, sì, negli ultimi trenta anni, abbiamo avuto una non cultura nella pubblica amministrazione, nella misura in cui all'amministratore arrivato nell'ente si fosse posto il problema di quanti sono i denari che dobbiamo spendere. spendere. Per questo motivo, riteniamo che la norma del 2 per cento non soltanto consentiva una elasticità nel divenire del funzionamento degli enti locali e dei Ministeri, ma era anche virtuosa e pedagogicamente valida perché cominciava ad istruire gli amministratori locali e centrali ad una logica che non fosse dello spendere quanto più possibile. Però, abbiamo avuto modo anche di vedere in questo provvedimento una disattenzione totale; anzi, un'azione di rivolgimento rispetto allo Statuto del contribuente. Chi, come me e come molti di voi, è stato padre dello Statuto del contribuente, sa quanto abbiamo creduto in questo strumento come soluzione anche per mettere lo Stato nelle condizioni di essere patrio Governo ed il contribuente di essere cittadino. Ma voi calpestandolo, con questo provvedimento, ci mettete nelle condizioni di dover ricominciare a fare una sorta di pedagogia per convincere il contribuente a considerarsi cittadino. Ci auguriamo che presto questo Governo smetta la sua funzione perché ci dispiacerebbe oltremodo che i danni notevoli che si procurano con una esagerata pressione fiscale, con una disattenzione notevole alla spesa per investimento, ci portino verso una Italia che non è quella che gli italiani vogliono; non è quella che, con manifestazioni in tutti gli ambiti, si sta dichiarando; non è quella che certamente voleva chi è venuto prima di noi, né vogliono coloro che verranno dopo di noi.

il decreto è uno degli elementi della manovra finanziaria per il 2007: è difficile e forse neppure utile discuterne facendo astrazione dal resto della manovra. Non è certo la prima volta che una legge finanziaria è accompagnata (all'inizio del suo viaggio) e preceduta (alla fine) da un decreto prevalentemente fiscale. E non è la prima volta che un decreto fiscale contiene anche norme ordinamentali. Peraltro, nei suoi effetti economici sui saldi di bilancio, la norma in oggetto ha disposizioni prevalentemente sul lato delle entrate, con effetti sull'indebitamento netto di 3.972 miliardi nel 2007, di 3.625 miliardi nel 2008 e di 3.844 miliardi nel 2009. Questa previsione di entrate, insieme alle disposizioni della finanziaria, ha ingenerato in molti autorevoli commentatori la preoccupazione che la manovra possa tarpare le ali ad una ripresa economica reale, ma non impetuosa, e - parrebbe - non in fase di accelerazione. La preoccupazione è accentuata dalla recente frenata di altre economie, come quella francese ed americana. Nel corso della discussione in Commissione l'opposizione ha ripreso, con serietà e dovizia di argomenti, queste preoccupazioni. Pur non nascondendomi che il pericolo c'è, mi preme sottolineare alcune circostanze che lo rendono, a mio avviso, meno incombente di quanto non si affermi spesso. Sono considerazioni che riguardano sia il decreto in sé, sia la manovra nel suo complesso. Per stimare gli effetti sull'economia reale non è alle entrate alla voce «saldo netto da finanziare» che si deve guardare, ma a quelle, assai inferiori, di circa 1,6 miliardi, alla voce «indebitamento netto»: solo queste sono, o meglio saranno «vere», non soltanto giuridico-finanziarie. Non devono essere prese in considerazione le entrate di cui ai commi 71 e 72 relativi alle auto aziendali: a queste entrate fanno riscontro, in analoga misura, il minor gettito IVA conseguente alla riconosciuta deducibilità dell'IVA autoveicoli in seguito alla nota sentenza comunitaria, con effetto neutro sul complesso dell'economia reale. Si badi che ho parlato di minor gettito IVA, non di restituzione IVA non dedotta negli anni pregressi. Si è svolto nel corso dell'estate un dibattito sull'opportunità di un rientro rapido del debito pubblico, sostenendosi da parte di alcuni che un rientro rapido avrebbe effetti recessivi o non espansivi. Senza entrare nel merito della discussione (che peraltro non è certamente solo accademica, anche se condotta da accademici), rilevo come la manovra, rispetto al DPEF, sia spostata verso una permanenza di un debito elevato, almeno per due aspetti. come dimostra la Nota di aggiornamento al DPEF, il rimborso conseguente alla sentenza IVA (rimborso, non riequilibrio degli effetti) avverrà a debito. Infatti, la tabella 1 a pagina 3, quinta riga, registra previsionalmente fino al 2011 una discrepanza di 1,1 punti percentuali del debito pubblico sul PIL tra debito e debito al netto della sentenza IVA. come alcuni osservatori internazionali hanno fatto osservare, al di là delle configurazioni in sede di contabilità nazionale e comunitaria, lo spostamento di parte del TFR all'INPS si configura sul piano dell'economia sostanziale come un aumento di debito. Si badi che questa non è una critica al provvedimento, tanto meno una condivisione dell'opinione favorevole al mantenimento del debito pubblico attuale. Vorrei solo criticare le opinioni di quanti non vedono i possibili effetti espansivi di questa manovra del dibattito in Commissione l'opposizione ha sottolineato, non senza ironia, il gran numero di correzioni che il decreto in questione contiene al decreto Bersani-Visco: ma non è forse prova di saggezza e modestia riconoscere e correggere i propri errori? Si è sottolineato come soprattutto le norme ordinamentali non avrebbero carattere di urgenza, ma molte, se non tutte, lo hanno, basti pensare, per fare un esempio di non grande rilievo almeno per i non addetti ai lavori, alla norma sul compenso per il prestito librario: espunta dalla finanziaria, per intervento della Presidenza della Camera, è stata inserita nel decreto per porre riparo ad una inadempienza dell'Italia, risalente sì nel tempo, ma acuita da una recentissima sentenza di condanna in sede comunitaria. Come è noto, e ne ha parlato il senatore Morgando, anche per rispettare i tempi complessivi della manovra, la maggioranza ha deciso di non proporre emendamenti e si è espressa in Commissione contro quelli dell'opposizione. Si sono presentati però degli ordini del giorno, discussi a fondo, anche con parte dell'opposizione. Alcuni di questi ordini del giorno sono stati accolti dal Governo, altri sono stati votati senza il consenso del Governo. La materia è pienamente documentata, come è ovvio, negli atti parlamentari. La speranza è che parte dei contenuti degli ordini del giorno possano trovare spazio in prossimi provvedimenti legislativi, a cominciare dalla legge finanziaria stessa. Ricorderò alcuni degli impegni

una norma che vincoli a diminuzione di pressione fiscale l'eventuale maggior gettito tributario sostanzialmente, ascrivibile agli sperati successi, anche indiretti, dei provvedimenti antievasivi, antielusivi o comunque tendenti a recuperare base imponibile. l'impegno a riconsiderare, sulla base delle decisioni di Bruxelles in tema di detraibilità limitata dell'IVA degli autoveicoli, le norme della non deducibilità dal reddito delle spese per autoveicoli. le norme che impegnano il Governo a riconsiderare, anche alla luce di eventuali pronunciamenti europei (o per prevenire tali pronunciamenti), la normativa sulle concessioni autostradali. II Governo ha soltanto parzialmente accolto un ordine del giorno articolato, che utilizzava anche proposte avanzate dall'opposizione, in tema di imposta di successione. È stato accolto dal Governo il chiarimento che il valore degli immobili è quello cosiddetto catastale e non quello di mercato; non è stata accolta la richiesta di escludere oneri spesso insostenibili per aziende piccole o medie, al momento del passaggio *mortis causa* (o in vista di tale passaggio), pur nella consapevolezza che la disciplina vigente nel 2001, riattualizzata dal decreto in esame, esclude l'avviamento dall'attivo aziendale. Giungo alla conclusione: è un provvedimento ampio, organico e viene inserito in una manovra a sua volta organica. È vero che ci sono molte critiche nel Paese e molte manifestazioni contrarie, l'unico organo che non ha reagito negativamente a questa manovra è la Borsa italiana che è ai massimi dall'inizio del 2000. Questa mi sembra una circostanza che varrebbe la pena sottolineare, a meno che forse in Borsa non ci siano i poveri che ridono. Si sono criticati molti aspetti: sono passate sotto silenzio tante soluzioni felici, come la riforma del catasto terreni, collegata proceduralmente con la richiesta di contributi comunitari, un provvedimento di notevole impatto economico, a partire dal 2008, che non ha suscitato proteste forse perché riconosciuto equo. I giornali e le televisioni parlano molto più spesso del Libano che della Svizzera: nel decreto al nostro esame c'è tanta Svizzera e pochissimo Libano. Approviamolo, per la tanta, tantissima parte buona che in esso c'è e di cui ci si vuole dimenticare.

Signor Presidente, colleghi senatori, il decreto al nostro esame è parte integrante della manovra finanziaria in quanto si configura, è stato già detto nel dibattito, come significativa fonte di copertura della legge finanziaria stessa, per un ammontare pari a 6.900 milioni di euro. Peraltro, non è la prima volta

ciò ha costituito una prassi usuale, fino ad arrivare, in alcuni casi, ad adottare decreti‑legge collegati alla legge finanziaria,

deve lavorare per fare un passo avanti rispetto al DPEF, soprattutto sulla linea della necessaria contestualità tra risanamento, equità e sviluppo. Il decreto in esame, infatti, contiene, in prevalenza, norme di carattere fiscale e di riorganizzazione della pubblica amministrazione che sono urgenti sia perché, come ho detto all'inizio, va coperta la finanziaria (quasi sette miliardi di euro) e sia perché è necessario che alcuni effetti economici importanti possano partire dal 1° gennaio 2007. 2007. Lo voglio dire con franchezza a qualche collega che denuncia l'eccessiva influenza di Rifondazione Comunista o della cosiddetta sinistra radicale su questo provvedimento e, più in generale, sulla materia finanziaria: noi avremmo preferito un testo più corposo, rispetto a quello presentato dal Governo, ad esempio sul tema della nuova normativa della tassazione delle rendite finanziarie che, a nostro avviso, avrebbe trovato migliore collocazione in questa sede, piuttosto che in un disegno di legge presentato come collegato alla finanziaria (atto Camera n. con un miliardo di copertura per il 2007 e due miliardi per il 2008 e il 2009); avremmo preferito discuterne in questo seno e non come delega al Governo come collegato alla finanziaria. le misure previste sono importanti per continuare la lotta all'evasione fiscale, già iniziata con il decreto Bersani-Visco, come ha sottolineato molto opportunamente il collega Morgando. In particolare, è previsto il potenziamento degli apparati di controllo, sia contro l'evasione fiscale e contributiva che contro il lavoro nero. Su questo aspetto abbiamo presentato un ordine del giorno che ritengo molto importante, in cui si invita il Governo a valutare l'opportunità di adottare, sin dalla prossima legge finanziaria, interventi volti a integrare l'organico delle amministrazioni centrali e periferiche della pubblica amministrazione che risultino sotto organico, con priorità quei settori direttamente impegnati nelle attività di controllo, accertamento e riscossione dei tributi e del contrasto all'evasione fiscale e contributiva, nell'attività di ispezione e di vigilanza della sicurezza nel lavoro, valutando, a tal fine, la possibilità di attingere a graduatorie di idonei di concorsi pubblici già espletati.

vogliono segnare un rapporto nuovo tra risanamento, quindi rigore, e sviluppo. Desidero soffermarmi molto brevemente sulle misure a favore dell'efficienza energetica, nonché della sostenibilità ambientale, che stabiliscono un regime di agevolazioni al fine della diffusione dei mezzi di trasporto ad alta sostenibilità ambientale, misure a favore dello sviluppo, che dispongono la sospensione dell'applicazione degli strumenti di programmazione negoziata della nuova disciplina sui meccanismi di concessione degli incentivi alle imprese introdotti dal cosiddetto decreto sulla competitività. di un segnale importante di discontinuità. Sono, di conseguenza, revocate e riesaminate dal Ministero dello sviluppo economico le proposte di contratti di programma approvate dal CIPE e le relative risorse, unitamente a quelle derivanti dalla ritardata attivazione del fondo rotativo per il sostegno alle imprese. C'è una destinazione delle risorse che avanzano alla copertura degli oneri derivanti dai contratti di programma rimasti privi di copertura: si tratta di una misura importante per il Mezzogiorno. le disposizioni in materia di lavoro - a cui ho già accennato riferendomi all'ordine del giorno - sono finalizzare a stabilire e rafforzare il ruolo della commissione centrale di coordinamento delle attività di vigilanza ispettiva che diviene sede permanente di elaborazione di obiettivi strategici e prioritari dell'attività, nonché di monitoraggio di interventi attuati. Viene anche modificata la composizione di tale commissione al fine di valorizzare nella stessa il ruolo dell'Arma dei carabinieri, introducendo analoghe modifiche alla composizione delle commissioni regionali e provinciali. Nel settore lavoristico sono

pongono un problema di disciplina di contributi e provvidenze alle imprese editrici di quotidiani e di periodici, nonché a quelle radiofoniche e televisive, con un riordino dei criteri di calcolo dei contributi spettanti, dei costi ammissibili, dei tempi e delle modalità di istruttoria, di concessione e di erogazione, nonché dei controlli da effettuare. Siamo d'accordo e tuttavia

è stato soppresso l'articolo 26, come inizialmente era stato formulato, ribadendo in questo modo il carattere di diritto soggettivo dei contributi all'editoria *no profit*. Questa scelta è essenziale, lo dico anche ai colleghi dell'opposizione, per la sopravvivenza di testate storiche (penso a «il manifesto», al «Secolo d'Italia», ad «Europa», ecc.) e più in generale dei giornali di partito, che rappresentano voci importanti per lo sviluppo del pluralismo, in particolare per le testate autogestite o gestite da cooperative o da soggetti *no profit*. Ebbene, nell'ordine del giorno si chiedeva al Governo uno stanziamento triennale, non solo annuale, dei fondi necessari a coprire il fabbisogno di spesa dei contributi diretti e previsti dalla legge n. 250 del 1990 e a contenere la riduzione dei contributi per le agenzie di stampa, per le imprese di radiodiffusione dall'80 al 70 per cento e non al 60 per cento, come previsto invece da questo decreto-legge.

Vorrei concludere con una battuta, senza scomodare importanti economisti di questo secolo. Il rilancio dei consumi interni che è la conseguenza immediata di una politica nuova, avviata anche con il decreto Bersani-Visco, è un rilancio di quei consumi alimentati, ad esempio, da quei soggetti deboli e poveri che, con questa manovra finanziaria e anche con questo decreto, troveranno maggiori condizioni per vivere e avere un reddito. Ecco perché, invece di demonizzare la cultura dei diritti, bisogna valorizzare l'idea di uno Stato moderno dove ognuno partecipa allo sviluppo ma dove, soprattutto, ognuno è messo nelle condizioni di partecipare a questo sviluppo.

Prendo atto, per l'ennesima volta, che il Ministro considera forse più attraente interloquire in televisione con Fabio Fazio piuttosto che con i senatori. Vorrei ricordare al Ministro, per il suo tramite, che la nostra è tuttora una Repubblica parlamentare

Dunque, il Governo dovrebbe onorare qualche volta quelle parole con i fatti e non abbandonare quest'Aula all'assenza permanente di un suo Mi rendo conto di come il ministro Padoa-Schioppa non abbia molta confidenza con il sistema democratico e della rappresentanza. Egli ha percorso la carriera di alto burocrate e non ha avuto occasione di confrontarsi con il corpo elettorale. Proprio per questa ragione, però, dovrebbe avere maggior rispetto e sentire maggiormente il dovere di confrontarsi con chi il popolo lo rappresenta. Signor Presidente,dovrei chiederle per questo di interrompere la seduta in attesa che arrivi il Ministro. Mi limito ad invocare la sua sensibilità perché manifesti al Ministro il disagio del Senato nel non averlo mai visto partecipe dei lavori su importanti provvedimenti di

di farsi interprete di queste mie parole nei confronti del Ministro e attendo da lei una risposta al riguardo. Veniamo al provvedimento in esame oggi.

ma che il Presidente del Consiglio, il ministro Padoa-Schioppa, il vice ministro Visco e tutti gli altri membri del Governo continuano a propalare propagandisticamente, nel tentativo di avvelenare il dibattito politico e le opinioni degli italiani.

riguarda proprio l'estensione della base imponibile sottratta al prelievo fiscale contributivo. E, fin qui, *nulla quaestio*: è opinione comune consolidata che ampia parte della nostra economia sia sommersa. Dove nasce il presupposto di malafede? Nasce quando il Ministro sostiene che nella scorsa legislatura si sarebbe verificata una riduzione del gettito delle entrate tributarie correnti in rapporto al PIL - fatto che si è effettivamente verificato prevalentemente per l'erosione della base imponibile, in conseguenza di condoni e sanatorie fiscali e non, invece, della riduzione delle aliquote e del recupero, in realtà, di base imponibile.

per riflettere il positivo andamento del gettito nei primi otto mesi dell'anno. In particolare, occorre notare che nel periodo gennaio-agosto 2006, l'IRE ha registrato una crescita del 6,4 per cento rispetto allo stesso periodo del 2005, l'IRES è aumentata del 20,2 per cento e l'IVA è cresciuta del 9,3 per cento. Alla luce di tali andamenti, le stime di preconsuntivo per il 2006, in termini di contabilità nazionale, sono state riviste al rialzo di 5,9 miliardi rispetto al DPEF, con una crescita del 7,4 per cento rispetto al 2005. È evidente ad tutti - e a tutti coloro che non siano in malafede

ha formulato la propria nuova curva delle stesse ed una serie di ulteriori provvedimenti, l'aumento del gettito non può che attribuirsi all'ampliamento della base imponibile, conseguenza naturale della riduzione delle aliquote e, in parte, anche dei condoni. condoni. Sui condoni, su cui si fa molto moralismo, si deve spendere anche qualche parola di verità: bisogna abbandonare quella idolatria delle tasse di cui il vice ministro Visco è il più accanito custode e sostenitore. avviso, infatti, in presenza di un'aspettativa di condono, aumenta l'inclinazione ad evadere il fisco: il contribuente, in altre parole, sarebbe incentivato ad evadere oggi nella speranza e nell'attesa di un condono fiscale domani. È un'affermazione che non corrisponde affatto ai comportamenti reali dei contribuenti, siano essi cittadini o imprese, e che può essere pronunciata solo da chi non ha alcuna confidenza con il mondo del lavoro. I contribuenti, se evadono, lo fanno perché l'impatto del fisco, oggi, sulla loro attività è tale da minimizzare il loro reddito o, talvolta, da rendere inutile il loro lavoro. Voglio avvalermi di un esempio concreto: mi riferisco ad un fatto che mi è accaduto proprio ieri.

è probabile che il oltre il 40 per cento (più di 360 euro) finirà in tasse nelle tasche dello Stato. In totale, circa 1.000 euro, su 1.500 euro di una transazione, sono finiti ieri nelle casse dello Stato e solo 500 euro hanno ripagato dell'attività di quel notaio e di quei collaboratori. È questo un sistema fiscale accettabile? Si può stigmatizzare chi cerca in qualche modo di sottrarsi ad esso? Credo che non abbiamo,

contro l'azione del nostro Governo e contro i condoni a cui hanno aderito tanti, ivi comprese le società, credo, del Presidente del Consiglio, oltre che i principali organi di stampa dei partiti allora di opposizione, oggi di maggioranza, di cui parlava prima il collega Tecce.

e nel 2003 - se non ricordo male - ho aderito al condono, pagando quello che si doveva per i dieci anni precedenti e pagando il canone per quell'anno. Da allora sono costretto, anche se non volessi, a pagare regolarmente il canone, perché da telespettatore sommerso sono emerso, sono nuova base imponibile che si è allargata. Questo è l'effetto di quei condoni e non l'incentivo all'evasione. Dove sta, invece, l'incentivo all'evasione, signor Presidente? Esattamente nella strada che sta seguendo il Governo; la strategia fiscale di questo Governo si fonda su decine di misure occhiute che avrebbero la pretesa di aumentare la penetrazione dei controlli e che rappresentano, invece, un inutile aggravio di costi per le imprese e un potentissimo incentivo ad evadere e a scendere nell'economia sommersa. nell'economia sommersa. Si inabisseranno nell'economia sommersa le piccole imprese gravate da burocrazia rinnovata e inutile, come era stato dimostrato, come l'elenco clienti e fornitori. Tutto questo ha un costo per le imprese; tutto questo porta le imprese ad avere costi amministrativi e burocratici maggiori che si rifletteranno sulla loro capacità competitiva non sono pochi i piccoli e piccolissimi imprenditori che stanno dicendo che vogliono liquidare l'impresa per decidere di lavorare nel sommerso. Così come si inabisseranno definitivamente nell'economia sommersa tutti quegli artigiani e professionisti che non potranno più regolare legalmente le loro transazioni in moneta contante. L'ansia che ha colto il Governo sulla tracciabilità dei pagamenti, per la quale si esclude progressivamente nel tempo l'uso della moneta fisica, oltre a violare il presupposto per cui viene emessa la moneta; sulla moneta c'è scritto pagabile a vista al portatore e la legge istituiva della lira... PRESIDENTE. Senatore Stracquadanio, bisogna che termini, perché ha già avuto due minuti in più sottratti al senatore Ciccanti.

oltre a violare il presupposto della moneta fisica, porterà a milioni di transazioni non registrate. Altri dovrebbero essere i provvedimenti di contrasto all'evasione fiscale: ridurre l'aliquota per renderla meno conveniente e introdurre il contrasto di interessi tra soggetti in economia. Se posso dedurre in parte le spese che sostengo, chiederò che vengano fatturate; ne abbiamo avuto un esempio efficiente nel campo dell'edilizia dove la deducibilità fiscale delle spese di ristrutturazione, che è andata dal 36 al 41 per cento, ha fatto emergere un'amplissima base imponibile. Non mi illudo, tuttavia, che queste misure possano essere fatte proprie anche da questo Governo. Questo Governo ama le tasse e ne distribuisce in quantità. Dunque, abbiamo solo un'esigenza: sperare che vada a casa al più presto. Per questo, signor Presidente, colleghi, il prossimo 2 dicembre sfileremo pacificamente e serenamente in centinaia di migliaia - speriamo in milioni - per le vie di Roma, al fine di far comprendere al Governo che la sua ora è venuta, che gli italiani, oltre il 60 per cento, dicono i sondaggi, vogliono che vada a casa. Stracquadanio, per quanto riguarda il primo problema che ha posto nel suo intervento, quello della presenza del Governo, non devo ricordare a lei, che è un esperto parlamentare,

Il risanamento finanziario ed una politica per lo sviluppo sono gli elementi caratterizzanti dell'attuale dibattito politico e, di conseguenza, anche dei provvedimenti di ordine finanziario che il Parlamento si appresta a definire nella rituale legislazione di fine anno. Il tema delle infrastrutture è fortemente caratterizzato da ambedue gli aspetti della questione. La disponibilità di risorse è limitata anche in conseguenza del lungo periodo di difficoltà economiche che ha caratterizzato l'intero contesto europeo in questi ultimi anni rispetto ad altre parti del mondo. Per questo, i già considerevoli ritardi nella realizzazione delle infrastrutture si sono ulteriormente amplificati, creando strozzature e precarietà nei collegamenti, che rischiano di limitare fortemente la ripresa economica. Oltre ad una scarsità di risorse, il tema delle infrastrutture ha risentito di una differente visione tra i due schieramenti politici nazionali. Queste motivazioni, che di solito sono basate su criteri ideologici più che economici, hanno finito col condizionare, spesso sotto la spinta di gruppi ristretti, decisioni fondamentali per promuovere lo sviluppo di interi contesti territoriali. Ne è derivato un quadro nazionale infrastrutturale decisamente carente ed inadeguato a supportare i contesti economici attuali e che rende impossibili o eccessivamente onerose le naturali esigenze di crescita e di sviluppo. Un problema che investe l'intero territorio nazionale (il Nord come il con situazioni di grave difficoltà o addirittura di emergenza in alcuni contesti territoriali definiti. Indubbiamente, le problematiche ambientali vanno tenute nella giusta e doverosa considerazione, ma la strumentazione e la legislazione di tutela, correttamente applicate, possono agevolmente consentire, grazie anche all'evoluzione tecnologica, lo sviluppo sostenibile. In tale direzione va fatto uno sforzo *bipartisan* che consenta di affrontare tali temi con più concretezza e minori condizionamenti teorici, al fine di maturare in maniera condivisa progetti e decisioni per la cui attuazione operativa sono necessari lunghi periodi. La programmazione necessariamente pluriennale e l'individuazione delle priorità vanno in qualche modo tutelate dal naturale ed ordinario alternarsi degli schieramenti politici alla guida del Paese. Ciò è possibile solo se in tali contesti si assumono decisioni convergenti a fronte dei lunghi tempi di realizzazione. In caso contrario, si rischia di distruggere ricchezza più che promuovere crescita economica e sociale. Molti aspetti si possono considerare sostanzialmente acquisiti: l'importanza sempre maggiore dei collegamenti marittimi (le cosiddette autostrade del mare); la necessità di una maggiore incidenza percentuale del trasporto ferroviario, soprattutto per le merci; l'adeguamento indispensabile di molte direttrici viarie come nuove realizzazioni per assorbire flussi crescenti di mobilità. Il tutto in un quadro di integrazione e di interconnessione come di consentita flessibilità. Parimenti, la rete infrastrutturale ha oggi una definizione che travalica gli angusti confini nazionali e trova un definitivo riferimento nel contesto europeo ed anche extraeuropeo, a tutti i livelli, compreso il trasporto aereo. Si pensi alle forti difficoltà in cui si dibatte l'aviazione civile di bandiera in Italia e all'ancora irrisolto dilemma tra Malpensa e Fiumicino, che sta penalizzando in maniera quasi irreversibile non solo l'Alitalia, ma anche il traffico aereo nazionale a vantaggio di quello mancanza di risorse quindi, ma spesso anche decisioni errate o addirittura incapacità di prendere decisioni, a fronte di interessi contrastanti, con danni sempre più gravi per l'intero sistema Paese. La stessa disponibilità di risorse economiche a volte non è adeguatamente verificata in funzione della strumentazione finanziaria disponibile, anche innovativa, come la finanza di progetto. D'altronde, è necessario che all'opinione pubblica venga trasmesso un corretto messaggio: sarà sempre più difficile garantire servizi gratuiti a carico della fiscalità generale e sempre più spesso opere e servizi saranno disponibili solo attraverso procedure di autofinanziamento a carico degli stessi fruitori. Il tutto in un quadro economico di compatibilità e sostenibilità. Un discorso che vale per la circolazione e per la sosta nei centri urbani, come è sempre più verificabile nelle nostre città, ma anche, ormai, per tutte le esigenze di mobilità delle persone e di trasporto delle merci.

La storica e ricorrente difficoltà a rendere economicamente equilibrata la gestione del servizio ferroviario, come il rapporto auto/abitanti, in Italia ormai ai vertici delle statistiche mondiali, sono dati di fatto dai quali sarebbe solo illusorio prescindere. Parimenti le intese a livello europeo non possono essere disattese ed i progetti in fase avanzata di sviluppo e realizzazione non possono essere bloccati, se non a prezzo di costi rilevanti. Vanno portati quindi avanti e conclusi i progetti già avviati o programmati, nella scala di priorità definita e con la massima accortezza nei confronti degli impegni assunti a livello internazionale (dal corridoio ferroviario ad alta velocità trasversale nel Nord d'Italia ai corridoi viari europei dal Nord al Mediterraneo), utilizzando le risorse disponibili ed attivando procedure specifiche anche innovative, senza fughe all'indietro o ricerca di giustificazioni più formali che sostanziali. In conclusione, desidero far riferimento ad una situazione specifica inerente il corridoio Berlino-Palermo come esempio della necessità di avere una visione, non più localistica dell'intervento, ma di respiro sopranazionale.

con gravi implicazioni sull'economia e sulla stessa sicurezza delle popolazioni interessate. Per questo motivo, nei giorni scorsi le Commissioni 5a (Bilancio) e 6a (Finanze) del Senato hanno approvato, con voto unanime, il seguente ordine del giorno: «Il Senato in sede di esame del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, stante quanto previsto dall'articolo 2 comma 92, considerato che nell'ambito dei sistemi stradali e autostradali del Corridoio

al fine di razionalizzare e migliorare i collegamenti viari tra Campania e Lazio, che soffrono del restringimento della sezione a sud della provincia di Latina, impegna il Governo: a verificare con la Regione Lazio possibili modifiche o integrazioni degli accordi definiti tra Regione e Stato

La strada serve per collegare il Sud con il Nord, perché ci sono migliaia di autotreni che vanno al Sud come al Nord, c'è un centro ortofrutticolo a Fondi, che è il più grande d'Europa,

Signor Presidente, tra le molte ragioni di condivisione della manovra economica predisposta dal Governo per conseguire il risanamento dei conti pubblici, sostenere lo sviluppo e garantire un profilo di equità nella ripartizione del peso della manovra stessa, uno degli elementi più qualificanti che costituisce un tratto peculiare proprio del decreto-legge di cui oggi si discute, è quello di aver posto come una priorità l'impegno nella lotta all'elusione e all'evasione fiscale. È un titolo di merito del Governo e della maggioranza aver avviato da subito in questa legislatura, già col decreto Bersani-Visco del giugno scorso, una serie di misure volte a rendere più incisiva l'azione di accertamento e di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale che oggi, con le norme previste dal decreto collegato alla finanziaria, vengono ulteriormente affinate e migliorate. Mi riferisco alle disposizioni per la riforma delle riscossioni, di cui si sentiva l'assoluta necessità e l'urgenza, a quelle per rafforzare l'Agenzia delle dogane e la Guardia di Finanza nei controlli contro la contraffazione e l'invasione delle merci che giungono nel nostro Paese in modo inappropriato, oltre che per il potenziamento delle attività degli agenti accertatori. Misure serie, che seppur generano incombenze che possono risultare forse anche un po' fastidiose, hanno giustificazione - e che giustificazione! - nel fine che si ripromettono di conseguire. La lotta all'elusione e all'evasione fiscale, infatti, oltre che un primario fatto di equità, è un fattore di modernizzazione e di sostegno alla competitività del nostro sistema economico e sociale: sociale: sono i Paesi che hanno meno diseguaglianze in termini di distribuzione del reddito quelli che producono di più e innovano maggiormente. La domanda che vorrei porre ai colleghi del centro-destra, che pure a parole dichiarano di condividere questo obbiettivo è la seguente: in che modo pensate si possa aggredire una dimensione di evasione che oscilla tra il 27 e il 48 per cento del PIL, al punto di far dire a qualificati studiosi che questa è - paradossalmente, è ovvio - una delle industrie trainanti del nostro sistema economico negli ultimi dieci anni? È un'iperbole amara, ovviamente, se solo si guarda a che prezzo tutto questo avviene (penso alla minore trasparenza dei mercati, penso al*vulnus* che si reca ai principi della concorrenza, all'iniquità del carico impositivo, che viene a gravare tutto e solo sui contribuenti leali ed onesti, siano essi cittadini, famiglie, imprese). Questa è un palla al piede alla modernizzazione del Paese, ed è una situazione non più sopportabile, un'anomalia che va estirpata. Per ciò, sinceramente, non mi convince la demonizzazione che viene fatta da parte della destra, anche in interventi sentiti in quest'Aula, delle misure di rafforzamento delle capacità di accertamento, ed è paradossale sostenere, come qualcuno anche stamattina, ed anche in Commissione, ha fatto, che applicare la linea Visco vorrebbe dire, nei fatti, agire per incentivare l'evasione fiscale, quasi a giustificare il ribellismo di contribuenti che si vorrebbero angariati. Non è proprio così, perché la politica delle misure leggere, degli ammiccamenti di complicità e di giustificazione, tramite condoni e sanatorie, noi l'abbiamo sperimentata, come filosofia, nei cinque anni di Governo del centro-destra, ed è stato il «tremontismo», e cioè una politica che poi ci ha consegnato un quadro poco edificante del Paese, quello di un Paese che è privatamente molto ricco e pubblicamente molto povero. Sia ben chiaro: in Italia esistono i poveri, ce ne sono anche troppi, l'11 per cento delle famiglie (7 milioni e mezzo di individui ) è in condizioni di povertà e ci sono anche tante famiglie che hanno redditi con cui si fatica a vivere e anche il fatto che il 90 per cento dei contribuenti sia al di sotto dei 40 mila euro ci dice di un Paese che che in questi anni si è impoverito, e in cui anche i ceti medi hanno subito un livellamento verso il basso. Ma per converso, di fronte a tutta questa situazione, il dato eclatante, che si è accentuato negli ultimi anni, è che esiste un 20 per cento di famiglie che ha accumulato redditi privati che sono ai livelli più alti sul piano europeo, redditi conseguiti magari con l'evasione e con l'elusione fiscale, ed è proprio questa accumulazione di ricchezza privata, non sempre visibile, che lascia povero il versante pubblico e impedisce di riequilibrare e redistribuire risorse, servizi, opportunità verso chi ne avrebbe invece dritto. Se si ragiona su come in questi anni ci sia stato un grande sviluppo della ricchezza finanziaria, con i grandi stipendi ai *manager*, lo *stock option*, allora come si può non apprezzare le misure di parificazione a livello europeo, di armonizzazione delle aliquote sulle rendite finanziarie rispetto ad altri tipi di redditi di risparmio? E come non vedere, nella campagna di propaganda che è stata scatenata contro la finanziaria tutta tasse, oltre che la strumentalità, anche il riflesso di una cultura, vorrei dire di una incultura, che tenacemente rispunta ogni volta che c'è dibattito su questi temi, e che il centro-destra ha la responsabilità di avere incentivato e di incentivare, e cioè il fatto che pagare le tasse è qualcosa di sbagliato? È chiaro che si può discutere sui livelli di tassazione, ma le regole occorre rispettarle ed il fisco, come cercano di fare questo decreto e le manovre della finanziaria, può essere una leva di redistribuzione importante, ma occorre che le tasse si paghino e le paghino tutti, altrimenti si finisce col colpire sempre e solo una parte, radicando una pesante ingiustizia e portando al limite, per quella parte che le paga, l'insostenibilità della pressione fiscale. Un altro merito del decreto che discutiamo è poi quello di avviare e concretizzare importanti riforme strutturali, da lungo tempo attese e rivendicate, mi riferisco in particolare alla questione del passaggio e del lavoro che coinvolge i Comuni a proposito del catasto: qui il trasferimento di una serie di competenze riveste un alto valore strategico al fine di riordinare il sistema degli estimi e di classamento degli immobili, con possibili riflessi, a parità di gettito, sul piano dell'equità nell'applicazione dell'ICI. Non condivido le profezie nefaste che qualche collega dell'opposizione ha svolto in Commissione e forse svolgerà anche in quest'Aula riguardo ad un sistema che rischierebbe di frammentarsi in ragione delle scelte discrezionali delle varie amministrazioni e che porterebbe inevitabilmente ad un aumento della pressione fiscale. In primo luogo, perché i parametri a cui ci si deve riferire tengono conto di dati censuali, dei tempi di costruzione, della morfologia dei tessuti urbani, delle previsioni di pianificazione territoriale, cioè tutti elementi certi e trasparenti, e poi perché dalla responsabilizzazione maggiore dei Comuni, com'è nello spirito del federalismo, può derivare una migliore valutazione della appropriatezza relativa di una classificazione e si possono praticare criteri molto più aderenti all'effettivo valore immobiliare, con indubbie ricadute di equità per i contribuenti e maggiori strumenti di governo nella gestione delle problematiche di sviluppo urbano. In questo modo, tra l'altro, si compie un passo nella direzione, dal mondo delle autonomie, di un riordino complessivo della tassazione sugli immobili da semplificare, alleggerire e ricondurre alla piena competenza degli enti locali come uno degli aspetti con cui sostanziare l'autonomia e il federalismo fiscale. Un approccio serio, quindi, e necessariamente processuale, tutt'altra cosa dalle suggestioni semplicistiche e, mi si permetta, demagogiche. Girando per Roma, la settimana scorsa, ho visto manifesti di Alleanza Nazionale a favore dell'abolizione dell'ICI sulla prima casa. Non ho niente contro questa proposta: in 25 anni non mi è mai capitato di incontrare un Sindaco che facesse a gara e fosse contento di applicare l'ICI - che, lo ricordo, fu data ai Comuni come cespite compensativo di trasferimenti unilateralmente soppressi dallo Stato e sul tema il centro-sinistra ha le carte in regola, perché fu proprio negli anni dal 1996 al 2001 che si tolse l'IRPEF sulla prima casa. Ma se si vuole *tout* *court* l'abolizione dell'ICI sulla prima casa, bisogna poi dire come si compensa quel gettito e, mi permetto di dire ai colleghi di Alleanza Nazionale, si potrebbe cominciare proprio con l'apprezzare le norme sul catasto contenute in questo decreto-legge, che permette proprio di operare anche in quella prospettiva, seppure gradualisticamente, consentendo di recuperare gettito che potrà anche essere orientato alla riduzione dei carichi sulla prima casa. Da ultimo, anche la critica che il centro-destra rivolge alla manovra, che sarebbe poco efficace e anzi sbagliata, perché non si muove sul duplice binomio della riduzione del prelievo fiscale complessivo e della contestuale riduzione della spesa corrente, è davvero poco convincente. Non solo perché viene da fonti - i colleghi del centro-destra - che nel quinquennio passato non hanno ridotto la pressione fiscale (che, anzi, nel 2006 cresce di un punto di PIL rispetto al 2001) e hanno lasciato crescere la spesa corrente del 2,7 per cento in un quinquennio, ma anche perché se si prende solo il metro della riduzione della spesa, guardando anche agli emendamenti che sono stati presentati e che l'Assemblea dovrà valutare, si avrebbero conseguenze pesantissime: il taglio del 90 per cento dei contributi in favore di enti, istituti e associazioni; pesanti riduzioni sulle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, dei servizi di trasporto urbano; penalizzazioni sul tema degli investimenti, sul volume degli investimenti pubblici e sui trasferimenti correnti alle imprese. Insomma, solo pochi esempi, ma utili a dare il senso di quali sarebbero le ricadute in termini sociali della politica dei soli tagli alla spesa ed è anche assai dubbio che misure di questo tipo (penso solo alla diminuzione del capitolo degli investimenti o al taglio del 90 per cento sui trasferimenti alle imprese) non avrebbero effetti depressivi sull'andamento della nostra economia. Per questo insieme di considerazioni, quindi, esprimiamo una convinta adesione e sostegno all'impostazione del decreto che oggi siamo chiamati a discutere ed approvare.

*(Ulivo)*. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, il decreto-legge in esame è uno dei provvedimenti che, unitamente ai disegni di legge di bilancio e finanziaria, compone la manovra finanziaria per l'anno 2007. Esso manifesta la sua coerenza con gli obiettivi perseguiti dalla politica economica del Governo, con particolare riferimento alla necessità che il nostro Stato rispetti i parametri fissati in sede comunitaria. Uno dei dati di base dai quali dobbiamo partire per comprendere le preoccupazioni di Bruxelles è costituito proprio dal monumentale debito pubblico ereditato dai Governi Berlusconi, che in Europa non ha pari (da solo, ne rappresenta "solo" il venti per cento) ed è tra i più elevati di tutto il mondo sviluppato. Ciò detto, è vero che stiamo uscendo faticosamente da un ciclo, nel quale abbiamo avuto il più basso tasso medio di crescita: lo 0,3 per cento. Solo nove Paesi, tra i 180 monitorati, sono riusciti a fare peggio della destra al Governo in questo Paese! Ma non basta. Il passato Esecutivo ha accumulato qualcosa come 15 milioni di euro di debito, ha di fatto azzerato il disavanzo primario, incrementato di due punti percentuali la spesa pubblica corrente e ha tagliato i finanziamenti per le infrastrutture. In questi giorni, peraltro, sono emersi nuovi debiti delle Ferrovie, in parte conosciuti, ma comparsi nella loro reale effettività da sotto il tappeto da dove erano stati abilmente nascosti negli anni precedenti. La destra si era impegnata - purtroppo solo a parole - con l'Europa a far rientrare, entro il 2007, il rapporto *deficit*/PIL al di sotto del 3 per cento. Ma chi sta onorando con i fatti questo gravoso impegno è questo Governo. E come se non bastasse, oggi dobbiamo anche sopportare le «grida manzoniane» di coloro che parlano di finanziaria "lacrime e sangue"! E' veramente sorprendente come, dalla gabbia degli imputati, oggi la destra pretenda di saltare, con un balzo rocambolesco, al banco degli accusatori!

Sul piano internazionale va, tuttavia, osservato che l'«ombra lunga» di una possibile, pesante crisi proveniente dal Nord-America si sta allungando sull'economia mondiale ed i recenti risultati delle elezioni di medio termine non lasceranno indifferenti i mercati e gli operatori finanziari. Nonostante questo scenario, le cose nel nostro Paese da qualche mese stanno lentamente migliorando. Secondo la Confindustria, la produzione industriale, fra l'ottobre del 2005 e l'ottobre del 2006, è cresciuta del 3,2 per cento: potremmo azzardare a definirlo un «piccolo *boom*», soprattutto se confrontiamo questi dati con gli «ansimanti» indicatori degli ultimi cinque La nostra crescita economica (all'interno di una ben maggiore crescita dell'area euro stimata, per l'anno in corso, intorno al 2,7 per cento) si sta avviando ai due punti percentuali, contro una previsione iniziale di appena l'1,6 Questo dato dovrebbe farci sperare per il prossimo biennio. Senza spingerci troppo in avanti, Governo e maggioranza potrebbero essere seduti sopra ad almeno 1.000 giorni di buona crescita; elemento questo che costituisce una piattaforma sulla quale si è via via andata edificando la legge finanziaria, di cui oggi esaminiamo il decreto-legge collegato. Mille giorni di buon vento nelle vele possono servire per fare molte cose, se non per cambiare il Paese, certamente per migliorarlo, e molto. Per questo è stato necessario concentrarci sulle priorità, senza alcuna volontà di rivincita ideologica, ma predisponendo le basi per una fuga in avanti verso quelle che saranno le grandi riforme da impostare. Tra gli interventi prioritari contenuti nel decreto-legge in esame, ne vorrei evidenziare soltanto alcuni, Presidente: la pervicace lotta all'evasione e all'elusione fiscale; misura, questa, della quale il Governatore della Banca d'Italia ha sottolineato la giustezza e l'opportunità, in una chiara prospettiva della riduzione della stessa pressione fiscale («pagare tutti per pagare meno»); azione che verrà condotta anche attraverso una complessa operazione di rimozione delle macerie accumulate dal precedente Governo, dal definitivo abbandono della scellerata politica dei condoni, nonché del potenziamento dell'Amministrazione finanziaria; le misure di rivisitazione catastale che contribuiranno ad un razionale riordino delle rendite degli enti locali. Sul punto l'Ulivo non condivide le preoccupazioni di una certa destra circa il presunto aumento indiscriminato delle rendite catastali per effetto del trasferimento ai comuni del prelievo delle relative competenze, dal momento che tale misura non accresce il prelievo fiscale ma, al contrario, razionalizza il sistema di estimi e classamento degli immobili; le norme sul trattamento tributario delle *stock option*, sull'aliquota dell'accisa sui prodotti petroliferi, sull'accelerazione in tema di incentivi alle imprese, sull'evoluzione normativa riguardante le le imposte e sulle successioni e donazioni. A tale proposito vorrei richiamare, in particolare, l'attenzione sul trattamento fiscale delle donazioni effettuate in favore delle ONLUS, nonché di soggetti operanti nel terzo settore; la rideterminazione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca, previsto dalla legge finanziaria per il 2005, e della quale il precedente Governo aveva volutamente ritardato l'attivazione per fare cassa; investimenti per le infrastrutture, tra le quali ANAS e Ferrovie, per le quali il passato Esecutivo, di nuovo, aveva azzerato le risorse. Il provvedimento in titolo dispiega a favore dell'ANAS tutta una serie di interessanti prospettive ispirate a princìpi di maggiore efficienza, controllo, trasparenza, nonché alla nuova disciplina relativa ai rapporti concessori sui quali anche bisognerà fare ulteriori aggiustamenti in norme future. Sul punto, durante l'*iter* dibattimentale in Commissione bilancio è stato fatto proprio un ordine del giorno, il quale punta a rendere più stringenti gli obblighi in capo ai concessionari in ordine agli investimenti, alle manutenzioni, nonché alla qualità dei servizi per gli utenti; il potenziamento infrastrutturale della Sicilia e delle aree limitrofe, atteso che si intende recuperare le risorse già stanziate per la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina, non più tra le opere nel programma del Governo; le misure nel settore dell'editoria e delle comunicazioni, ove si interviene in modo significativo al fine di dare un'impostazione moderna ed europea ed europea ad una materia particolarmente delicata, la quale, peraltro, sta vivendo da mesi una difficile vertenza tra editori e giornalisti. In questo comparto, le forze di Governo intendono perseguire lo snellimento delle procedure di erogazione e controllo; la crescita dell'efficienza, ma anche dell'occupazione e dell'innovazione. Anche su questo aspetto, durante l'*iter* dibattimentale in Commissioni bilancio e finanze riunite, è stato fatto proprio e accolto dal relatore un ordine del giorno, a firma dei senatori Tecce, Barbolini e del sottoscritto, con il quale si è rappresentata l'esigenza di una maggiore attenzione nei confronti della editoria *no profit* e delle imprese di radiodiffusione. A quanti oggi ci chiedono di più, rispondiamo che questa manovra di bilancio non è e non può essere «l'alfa e l'omega» del Governo: è solo il primo passo di scelte che si dispiegheranno nei prossimi quattro anni e mezzo. Chi ci accusa di dirigismo, dimentica in fretta le leggi di bilancio della destra, improntate ad una filosofia qualunquista e populista; si rifiuta scientemente di vedere che l'impianto dell'attuale finanziaria, e quindi del decreto-legge in esame, che ne costituisce parte integrante, si fonda, per un verso, su un'attenzione particolare al mercato e, per altro verso, su una maggiore sensibilità alle prospettive delle nuove generazioni. Come spiegare le scelte per un fìsco da una riduzione del cuneo fiscale a vantaggio di imprese e lavoratori? Come spiegare la lotta all'evasione e all'elusione fiscale? Come spiegare, infine, l'impegno sulla previdenza complementare? Questi molteplici interventi altro non sono che segmenti di riforme indirizzate ad un unica realtà sociale, economica e produttiva, di un Paese come il nostro, che solo ora sta uscendo timidamente da un lustro di sofferenza. Se la destra italiana fosse veramente liberale come si proclama non si schiererebbe a fianco di interessi corporativi che alzano barricate e oppongono resistenza ad oltranza ogni volta che si sentono sfiorati. Se fosse veramente liberale sarebbe d'accordo con la riforma del TFR, che altro non è che la riforma Maroni anticipata di un anno, ma che proprio il precedente Governo ha congelato, allorché danneggiava le assicurazioni, *rectius*, alcune assicurazioni. Tutte le volte che in questo Paese la politica veramente liberale colpisce la corporativizzazione, l'oligopolio, gli accordi di cartello, i contingentamenti, la burocratizzazione e punta seriamente verso la liberalizzazione dei mercati, risorge lo spirito guicciardiano: la tutela a oltranza del «particulare», che nulla ha a che spartire con una società capitalistica, moderna e innovativa. Il provvedimento in esame costituisce un pilastro fondamentale della più consistente e corposa legge finanziaria che sarà oggetto di successivo esame, e consente di conseguire, oltre che maggiori entrate e miglioramenti dei saldi, una significativa redistribuzione della ricchezza, anche attraverso una maggiore equità fiscale. Non saranno pochi i passi che dovremo percorrere, ma l'importante è tenere la rotta, signor Presidente, nella convinzione sottile, ma invincibile, che un modello di sviluppo coniugato ad un vero progresso sociale è possibile. Questo servirà a quella comunanza di aspirazioni e speranze che uniscono gli individui e ne fanno una collettività e che fanno di una collettività un sistema Paese. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, con il decreto Visco-Bersani di luglio è stato previsto di recuperare oltre 5 miliardi di euro di entrate evase o eluse. Con questo decreto e in parte con la finanziaria 2007 si propone il recupero di imposte evase o eluse per circa 8 miliardi di euro. Gli strumenti Gli strumenti posti in essere si concretizzano in due strategie: la prima è volta al rafforzamento dei poteri e dei mezzi dell'amministrazione finanziaria per l'accertamento; è volta all'ampliamento dei poteri del fisco, ossia dello Stato, nei riguardi del contribuente, creando una gigantesca anagrafe tributaria. Il presidente Casini ha detto a chiare note che l'evasione è un furto. Chi evade il pagamento delle imposte dovute ed usufruisce dei servizi e benefici pubblici finanziati da chi le imposte invece le paga, ruba sui sacrifici altrui e ruba futuro alle prossime generazioni. Due dati però ci dovrebbero aiutare a capire perché e come si deve affrontare il problema dell'evasione. Secondo l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, in Italia si stima vi sia un'evasione ed elusione di circa 200 miliardi di euro, per metà dovuta ad imprese, società e lavoratori autonomi, ma per metà dovuta anche a lavoratori dipendenti con doppio lavoro in nero e all'esercizio abusivo di attività produttive, commerciali e professionali, che alterano i prezzi e il mercato perché distorsivi della concorrenza. Secondo l'ISTAT e l'ISAE è stato calcolato un sommerso, cioè attività illegali, o se legali condotte senza rispettare le norme fiscali, pari a una percentuale che varia tra il 17 e il 23 per cento, rispetto a una media europea che si pone tra il 12 e il 15 C'è un Italia che vive sulle spalle degli altri, senza pagare pegno. C'è un altro dato su cui riflettere. Lo Stato registra una riscossione di tributi pari al 5 per cento rispetto a quelli accertati e sopporta un costo per gli adempimenti di tale riscossione intorno al 6 Non c'è proporzione, quindi, tra costi e benefici, sulla via della pretesa forzosa dei tributi. In questo decreto assume rilievo la maggiore attività di accertamento e contrasto alle evasioni fiscali in termini di IVA, IRPEF e IRES, che incidono sul saldo netto da finanziare, cioè sulla competenza, per circa 2 miliardi di euro, ma di cui si prevede un incasso, per il 2007, di soli 200 milioni di euro. Ci si rende conto di come siano diverse e lontane le strade del maggiore accertamento da quella dell'ampliamento della base imponibile, attraverso misure di emersione dell'elusione fiscale. Non c'è proporzione tra la poderosa «macchina da guerra» posta in essere con l'anagrafe tributaria! L'invadenza nella sfera della vita privata dell'operatore economico, conseguente all'attività di accertamento, i costi di adempimento richiesti agli intermediari finanziari e agli stessi operatori economici ed il risultato atteso, in termini di maggior gettito fiscale nelle casse dello Stato, non hanno proporzione. Su questo piano ci vogliamo confrontare, perché ci sono due culture politiche che si scontrano: innanzitutto quella di Visco e del centro-sinistra, che concepisce lo Stato come il grande Leviatano, sempre più tendente verso lo Stato etico, dirigista e di polizia che, occhiuto e malfidato, si attrezza con la logica del «Grande Fratello», perché il cittadino suddito sia sempre controllato, condizionato e subordinato, soprattutto se lavoratore autonomo autonomo o libero professionista, ovvero tosato bene, se imprenditore oppure operatore finanziario. C'è poi l'altra cultura di Governo, quella che ha ispirato la nostra azione negli anni scorsi, la cultura dello Stato liberale, di uno Stato amico del contribuente, di uno Stato che chiede ai produttori di ricchezza del Paese di esprimere solidarietà, secondo le regole del gioco degli interessi nazionali, degli accordi comunitari e internazionali, secondo i parametri politici ed etici della coesione sociale. È la logica della comunità nazionale, dove ciascuno è volontariamente chiamato ai doveri sociali per sentirsi parte dell'insieme: in tale logica riteniamo che il sistema Visco non funzioni. Non si governa il fisco con la paura e l'intimidazione, soprattutto verso chi le imposte le paga, le vuole pagare, ma ha difficoltà a pagarle, anche per colpa di una normativa ondivaga, complicata, contraddittoria e farraginosa. Prima di minacciare le manette, Visco metta ordine alle regole:

dallo Stato, come quella sulla irretroattività delle norme tributarie, prevista dallo Statuto del contribuente. Senatore

Non può esserci un commercialista per ogni contribuente: il nostro sistema di Governo del fisco, quello da Stato liberale, testimoniato dal centro-destra, ha portato all'emersione di una vasta massa di evasori ed elusori, con la logica della premialità, proprio attraverso i contestati condoni fiscali. Il nostro ragionamento è stato questo: contribuenti, sappiamo che molti di voi non pagano tutte le tasse e c'è addirittura chi non le paga affatto. Facciamo un patto: pagatele tutte e tutti. Se qualcuno nel passato ha fatto il furbo, gli garantiremo il perdono fiscale, così come il centro-sinistra ha fatto con l'indulto, che è un perdono giudiziale. Però attenzione: tutti coloro che non si autodenunceranno, saranno sottoposti ad accertamento e, se non saranno in regola con il fisco, saranno dolori.

perché tutti paghino le tasse, come già avviene per le visite mediche, per le ristrutturazioni edilizie e così come pensiamo debba essere per gli affitti delle abitazioni degli studenti universitari. È successo che nel 2005-2006 i due condoni, e senza considerare le entrate in conto capitale dei due condoni, che pure hanno fruttato allo Stato oltre 22 miliardi nel 2003 e quasi 12 miliardi di euro nel 2004, hanno determinato un aumento di gettito fiscale strutturale. Le entrate tributarie erariali rispetto al 2005 sono aumentate, sino al 30 settembre 2006, di 29,4 miliardi di introiti permanenti, così come riportato dal bollettino economico di questo mese della Banca d'Italia. È vero che una parte di queste imposte è dovuta alla crescita dal PIL dell'1,6 per cento, che ha comportato un maggior gettito fiscale, ma è altrettanto vero, però, che nel 2005 con crescita del PIL uguale a zero, il gettito delle imposte dirette è cresciuto rispetto al 2004 del 12,7 per cento e quello da imposte indirette dell'8,5 per cento, senza aumento della pressione fiscale, che è risultata del 40,6 per cento, inferiore quindi di un punto a quella del 2001 del centro-sinistra, che era pari al 41,6 per L'eredità che il Governo Prodi ha ricevuto dal centro-destra nel campo delle entrate permanenti è, dunque, buona e positiva, così come il Governo stesso ha riconosciuto nel DPEF. Ci sono altre questioni che non ci convincono più di altre in questo decreto-legge: la convenzione unica per le società concessionarie autostradali; la limitazione ai soli calciatori e non ad altri ben pagati miti dello spettacolo, della denuncia telematica dei contratti di sponsorizzazione; la palese violazione di domicilio da parte degli agenti della Riscossione Spa per il pignoramento dei crediti verso terzi senza il vaglio dell'autorità giudiziaria; la riduzione dei trasferimenti erariali ai Comuni in relazione all'aumento ICI dovuto alla rivalutazione del 40 per cento del moltiplicatore delle rendite catastali per i fabbricati di categoria B, riguardante ospedali privati, orfanotrofi, scuole private, case di assistenza ed altri servizi collettivi gestiti da cooperative ONLUS e istituti religiosi; l'aumento dell'accisa sul gasolio da trazione, perché si scarica sull'aumento dei carburanti delle auto diesel; l'aumento del bollo sui cinque milioni di motocicli da girare alle Regioni per un gettito previsto di oltre 83 milioni di euro, senza tenere conto che già le Regioni Veneto, Calabria, Campania, Marche, Lombardia e Piemonte adottano importi maggiorati sulla tariffa ordinaria; la cancellazione del ponte sullo Stretto di Messina, la perdita del 20 per cento del cofinanziamento europeo e i danni da risarcire alla società vincitrice dell'appalto; la riduzione dei contributi all'editoria e il mantenimento di sprechi e privilegi rispetto ad altri soggetti aventi diritto; lo *spoils system* operato contro ogni regola di Stato di diritto, con il licenziamento dei dirigenti non graditi politicamente, nonostante la documentata professionalità; l'ingiusta esclusione dei «fratelli» nella quota esente della imposta di successione e donazione, così come l'indifferenza dimostrata verso i trasferimenti intergenerazionali delle attività imprenditoriali che sono una risorsa per il Paese. Sono tutti argomenti per i quali abbiamo presentato emendamenti che tratteremo in tale sede di discussione, rafforzando così le ragioni del voto contrario dell'UDC a questo decreto-legge. In questo dissenso, però, siamo in buona compagnia, anche della maggioranza di centro-sinistra. Con 13 ordini del giorno, votati in tarda nottata, gli stessi membri delle Commissioni riunite V e VI hanno riscritto il decreto-legge, trasferendo tutti i cambiamenti alla prossima finanziaria. È onesto dire con noi: «Prodi?

ne è testimonianza lo stato di quest'Aula di questa mattina. Purtroppo, la discussione molto spesso verte sui dettagli anziché sulla politica economica per il Paese: quella di cui il Paese avrebbe bisogno e quella che in concreto viene seguita. Proverò ad attenermi a questo.

l'entità della manovra è adeguata rispetto a quello che ci serve? La quantità, direbbe un economista, è sempre la cosa più importante quando si parla delle politiche di bilancio e lo è particolarmente in Italia.

di quanto preleviamo dalle tasche dei contribuenti, anziché andare a pagare strade, asili e ferrovie, serve a pagare gli interessi su quel debito. Paghiamo più interessi perché abbiamo più debito ma anche perché, per ogni 100 euro di debito, paghiamo un interesse un po' più alto rispetto a questi altri Paesi. Quindi, il nostro problema di quantità riguarda alla fine quante strade, quante ferrovie, quanti asili nido siamo in grado di fare.

obiettivi. Dal 2001, ogni anno questo Paese ha annunciato un obiettivo senza riuscire a perseguirlo. I numeri di consuntivo erano diversi dagli obiettivi annunciati. Questo contribuisce a ridurre la credibilità del Paese e a farci pagare più interessi sul debito.

E' sufficiente a ritornare a ridurre il rapporto fra debito e ricchezza? E' sufficiente a raggiungere l'obiettivo da noi annunciato? La manovra, cioè, è adeguata perché il Paese ricominci a recuperare credibilità?

I problemi italiani sono lì: meno strade, meno ferrovie, meno asili nido derivano dal fatto che tale spesa è cresciuta molto in rapporto alla ricchezza per buona parte degli anni

ambiziosi, che i meccanismi di spesa sono difficili da piegare e che gli interventi di cui abbiamo necessità per piegare quella dinamica della spesa sono, come si suole dire, strutturali in quanto sostanzialmente intervengono sui meccanismi di lungo periodo che generano la crescita della spesa.

capacità di contribuire al miglioramento delle attuali condizioni dell'Italia. In particolare, si evidenzia un tentativo di contenere la spesa corrente per accrescere la spesa in conto capitale.

segnale. Una parte importante delle risorse reperite viene destinata a ridurre il costo del lavoro. Da lì può derivare una spinta alla crescita dell'economia e comunque alla crescita dell'occupazione. È un segnale buono di qualità della spesa.

tenterò, nella calma di quest'Aula, di mettere in evidenza le due proposte di politica economica che questa volta, più di altre volte, sono risultate chiare nella discussione e nell'esame parlamentare, cioè quella dell'opposizione e quella della maggioranza. Credo che il fatto che in modo evidente risultino due ricette di politica economica sia un bene: un bene per la nostra discussione e un bene, credo, anche per il Paese, per i cittadini che possono, in questo modo, formarsi meglio un'idea attorno alle cose che devono essere fatte per rimettere in movimento il nostro Paese. Faccio una premessa importante: questo provvedimento serve

aumenti di entrata derivanti dalla lotta all'evasione. È evidente che ciò produce un innalzamento della pressione fiscale: questo è obiettivamente e nei fatti. Questo decreto e la manovra finanziaria nel suo complesso produrranno effetti depressivi sull'economia nel 2007? Credo che senza problemi abbiamo già risposto, lo stesso Governo ha già risposto in sede di Documento di programmazione economico-finanziaria e in sede di finanziaria, perché nel 2007 si prevede una crescita del prodotto interno lordo di circa due decimali di punto in meno rispetto a quella che probabilmente si verificherà quest'anno. Ciò anche perché questa manovra, così rilevante dal punto di vista dell'entità, certamente avrà effetti anche di carattere depressivo sull'economia: questo credo che sia un dato assodato. Tuttavia, la discussione che dobbiamo fare è di altro tipo. Credo infatti che vi siano molti studi economici i quali dimostrano che gli effetti depressivi sull'economia sono minori se l'aumento delle entrate - come in questo caso - deriva dall'emersione di maggiore base imponibile. L'opposizione propone un'altra cosa: essa dice che bisogna diminuire le spese.

nell'entità proposta dall'opposizione. Ma ritengo anche che in questo momento attuare un'operazione drastica di riduzione delle spese delle spese produrrebbe un effetto depressivo sull'economia maggiore di quanto si produce attraverso un'azione di emersione di economia sommersa. Certo, diventa molto facile da parte mia ricordare - lo ha già fatto il senatore D'Amico - che nei cinque anni di governo della destra si è verificato l'esatto contrario rispetto a quanto si dice ora: infatti, nei cinque anni di governo della destra, la spesa corrente è aumentata di due punti e mezzo; si è, quindi, fatto il contrario di quanto si dice adesso.

Certamente, però, si inverte la tendenza che c'è stata in questi cinque anni: cioè, a fronte del fatto che per cinque anni la spesa corrente è cresciuta, con questa finanziaria, nonostante l'entità della manovra, si riduce la spesa corrente dello 0,1 Credo che questo sia significativo, perché è difficile fermare un treno in corsa, cioè la corsa dell'aumento della spesa corrente, tuttavia c'è questo segnale di inversione di tendenza. Al riguardo, credo che l'accordo con le Regioni sulla spesa sanitaria sia la dimostrazione dell'operazione che è stata fatta: c'è un aumento delle spese, ovviamente, perché la spesa sanitaria non si può comprimere e, tuttavia, questo avviene attraverso un processo di responsabilizzazione delle Regioni. Credo che questa sia la dimostrazione di come si possa, con misure adeguate, intervenire anche sul processo di contenimento della spesa corrente. C'è un aumento significativo delle entrate nei primi nove mesi. Prevalentemente crescono quelle

che ci sono più imposte dirette e crescono meno le entrate derivanti da quelle indirette, cioè da accise e tariffe, che sono quelle che incidono maggiormente sui redditi più bassi. bassi. L'opposizione, insieme alla riduzione delle spese, propone di ridurre il prelievo fiscale.

nel quale si dice che tutte le entrate superiori derivanti dalla lotta all'evasione fiscale dovranno essere finalizzate a ridurre la pressione fiscale e a rimodulare le aliquote. Credo che in questo momento non si possa fare altro.

Vedremo quanto aumenterà la pressione fiscale a seguito del provvedimento che stiamo esaminando. Però partiamo dal fatto che - ripeto - a politiche invariate, quelle realizzate dal centro-destra, la pressione fiscale è già aumentata.

La questione della lotta all'evasione è decisiva per l'azione di questo Governo, perché è un punto di forza della nostra azione, vi sono misure in discontinuità rispetto all'azione del precedente Governo. In Europa l'evasione

le misure devono essere varie, diverse, continuative e soprattutto efficaci. Queste misure hanno prodotto nel Paese alcune incomprensioni e anche alcune opposizioni, alcune di queste opposizioni sono comprensibili, su di esse occorre dialogare, occorre capirle, altre ritengo siano opposizioni di tipo corporativo, che devono essere respinte. Credo, come dicevo poc'anzi, che il Governo sarà più capito, nella sua azione di politica economica e di lotta all'evasione fiscale, se dirà in modo molto chiaro e limpido che tutte le maggiori entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale sono finalizzate a ridurre il carico fiscale, a ridurre le aliquote. Badate bene (a riguardo faccio un brevissimo inciso) c'è stata un'interpretazione circa il fatto che sono aumentate le entrate fiscali in questo scorcio di anno, un'interpretazione fornita da alcuni economisti, ma anche da una parte dell'opposizione, secondo la quale le entrate sono aumentate grazie ai condoni fiscali: in altre parole, facendo il condono si fa emergere base imponibile, la gente attraverso il condono si abituerebbe

quando interviene a un condono tombale che garantisce di sanare i contenziosi fiscali, i contenziosi amministrativi e i contenziosi penali, succede quello che si è verificato nel nostro Paese: si paga la prima rata e poi si torna in nero, e infatti le rate successive non vengono più

la violazione della *privacy* diventa un problema rilevantissimo nelle nostre società moderne, che poi è arrivato anche sulle prime pagine delle giornali a seguito delle cosiddette incursioni.

Gruppo. Come dicevo, ritengo che si debba evitare il proliferare delle cosiddette banche dati, anche perché alcuni dati sono già a disposizione si può accedere diversamente, non c'è bisogno ogni volta di creare una nuova banca dati, ma dobbiamo anche dire che oggettivamente sono proprio le nuove tecnologie informatiche che rendono in chiaro

chiedo scusa della battuta fatta durante l'intervento del senatore Ripamonti, con cui lo invitavo a concludere perché volevo intervenire ed essere così testimonianza vivente del presidio che l'opposizione porta all'arroganza di questa maggioranza che, nonostante i suoi attacchi alla cittadella della democrazia, trova imperitura resistenza in senatori che riescono a dire quanto il Governo stia sbagliando e quanto i colleghi della maggioranza stiano sbagliando nel difendere un provvedimento che è ingiusto nella sostanza, nella qualità e nella quantità. Il senatore D'Amico diceva che il provvedimento è giusto nella quantità. No: che sia ingiusto nella quantità non c'è bisogno che sia un senatore dell'opposizione a dirlo, perché lo dice il Governo oggi, nella sua apicalità più eccelsa, e cioè il suo Ministro del tesoro. Operiamo questo distinguo, perché oggi sappiamo che non esiste più un Ministro dell'economia, ma c'è un Ministro del tesoro - che è evidente non essere un «tesoro di Ministro» - e un ministro delle finanze, che è il ministro Visco. Essi hanno messo assieme una manovra finanziaria che non è assolutamente giusta dal punto di vista della quantità.

ti levo», come, ad esempio, nell'intervento nei confronti dell'intrapresa, alla quale con il cuneo fiscale si dà e poi si leva il TFR con una redistribuzione all'interno, con una manovra di una inutilità abissale. una osservazione che vorrei svolgere nei due o tre minuti che mi rimangono, è cioè che, di fatto, questa manovra si compone di una «grande finanziaria» e di una «piccola finanziaria», che giustamente sia la Camera che il Senato hanno giudicato essere un collegato e che giustamente i colleghi dicono essere un decreto collegato alla finanziaria e che ingiustamente il Governo invece

tutto un articolato che non ha niente di omogeneo, per cui finisce per essere un provvedimento di tanta spesa: basta citare l'intervento per il teatro Petruzzelli di Bari, che, se fosse stato inserito nella finanziaria, sarebbe stato espunto. Questo è un provvedimento fortemente contrario alla legge di contabilità e questo è importante perché, mentre il Governo fuori dall'Aula e i componenti della maggioranza in quest'Aula vengono a parlare della necessità di modificare la legge di contabilità, loro alla legge di contabilità hanno portato in questo momento la violenza più forte degli ultimi anni, cioè hanno prodotto una manovra finanziaria espungendo dalla legge finanziaria una parte evidente e portandola di fronte al Parlamento all'interno che non ha le motivazioni di urgenza come i decreti che sono stati presentati nelle legislature passate e che al suo interno contiene gran parte di misure non omogenee e una parte sostanziale di spese occultate, perché quelle sulle autostrade sono misure di spesa che non rendono assolutamente giustizia al fatto che il collegato dovrebbe essere omogeneo anche con il titolo perché dovrebbe recare disposizioni fiscali e non di spesa. Questo per dire che c'è una grandissima confusione e che il Governo in realtà si è messo alla ricerca per perigliosi sentieri di di riserve acquifere che potessero alimentare quelle cascate della spesa che fanno parte

non abbiamo la possibilità di cogliere il miglioramento dell'economia. Quindi, quella che in questo momento viene valutata come una diminuzione del PIL e che andrebbe ad essere scontata da un aumento della pressione fiscale,

una nuova finestra"). Comunico che il senatore Iorio ha inviato alla Presidenza la seguente lettera, in data 20 novembre 2006: «Caro Presidente, facendo seguito alla mia precedente nota del 10 novembre u.s., comunico che in data odierna, in esito alle elezioni amministrative svoltesi il 5 e 6 novembre scorsi, è avvenuta la mia proclamazione di eletto alla carica di Presidente della Regione Molise. Pertanto, rimetto le mie contestuali dimissioni dal mandato parlamentare di Senatore, a far data dal 20 novembre 2006. Nell'annoverare l'esercizio del mandato parlamentare tra le esperienze più positive e proficue del mio cammino politico, ringrazio per la disponibilità e lo spirito di collaborazione sempre riscontrati. *F.to*Michele Iorio». Trattandosi di un caso di incompatibilità - ai sensi dell'articolo 122, secondo comma, della Costituzione - il Senato non può che prenderne atto. Al senatore Michele Iorio, che cessa di far parte della nostra Assemblea, certo di interpretare il sentimento di tutti i colleghi, rivolgo un cordiale saluto e i migliori auguri di buon lavoro. Per consentire l'accertamento del candidato subentrante, autorizzo la Giunta delle elezioni a convocarsi sin d'ora.

con la quale il senatore Iorio, eletto in un modo che sottolinea il grande successo del centro-destra nell'ultima tornata elettorale, ha voluto rassegnare, come disposto dalla Costituzione, le sue dimissioni.